novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti***

Signora Presidente, desidero preliminarmente ringraziare la Commissione ambiente, il presidente D'Alì, il relatore Orsi e tutti i senatori e le senatrici intervenuti in Commissione, per i contributi forniti e per il lavoro svolto con spirito sereno e costruttivo.

più incisivo, per conseguire l'obiettivo principale che sta a tutti a cuore: avviare finalmente in Campania un corretto ciclo integrato dei rifiuti.

si è ritenuto valido e che non cambia, non essendo messo in discussione dagli eventi degli ultimi mesi. C'è stata una gestione non facile di alcune situazioni, penso ai problemi relativi

confermano le inchieste di questi giorni, ha dato anche la possibilità a organizzazioni criminali di innescare azioni violentissime. Vi è stato anche l'accumularsi di alcuni ritardi nelle procedure di realizzazione degli impianti. Questo provvedimento interviene con delle misure correttive contingenti, anche escludendo alcuni siti segnati dal disagio sociale, come Terzigno, dall'elenco delle discariche possibili, e con interventi strutturali

essenziali per rendere la Regione Campania autosufficiente nello smaltimento dei rifiuti. Credo vada ribadito anche in quest'Aula, perché è stato oggetto di interventi da parte di molti senatori, che c'è una profonda differenza fra la situazione attuale e quella di due anni fa; che c'è una grande differenza fra la gravissima emergenza sanitaria ed ambientale, che ha determinato pesantissimi danni a livello internazionale, e la situazione attuale, che registra una temporanea criticità causata da ritardi in un processo di normalizzazione del ciclo dei rifiuti che tutti dobbiamo volere. è stata ribadita in tanti interventi, di assimilare la situazione delle scorse settimane al dramma del 2008 posso comprendere che abbia valenza politica, che sia il tentativo di far passare l'idea che nulla è cambiato e che l'azione del Governo in verità non ha aggredito il problema, ma questo tentativo è smentito dai fatti: nel 2008 c'erano in strada 200.000 tonnellate di rifiuti, oggi quella criticità è stata superata. Napoli è è pulita e nei centri della Provincia restano meno di 4.500 tonnellate di rifiuti che nell'arco di giorni saranno eliminati. Il rapido superamento delle problematiche emerse nei mesi scorsi conferma che si trattava di problemi transitori, legati ad una difficoltà di gestione del sistema da parte degli enti locali della fase *post-*emergenziale. Direi che questa è una difficoltà comprensibile, se si considera che in Campania, in materia di rifiuti, si viene da 14 anni di commissariamento. La sfida che la comunità campana deve sostenere e vincere è quella di un ritorno all'ordinarietà, alle competenze del territorio, alla soluzione dei problemi dentro i confini della Regione. Il decreto-legge oggi in esame interviene per agevolare l'avvio, finalmente, in Campania di un ciclo corretto e moderno dei rifiuti attribuendo al Presidente della Regione il potere di nominare commissari straordinari per accelerare la realizzazione di impianti strategici ed essenziali e per individuare ulteriori siti da adibire a discarica. A questo riguardo, credo che una riflessione possa essere utilmente fatta in quest'Aula relativamente all'uso, per lo smaltimento di specifiche tipologie di rifiuti, delle cave dismesse, specie di quelle che sono transitate alla proprietà dello Stato. Credo che questa misura potrebbe rappresentare un segnale di grande utilità in questa fase di transizione, in un territorio in cui l'individuazione di aree da adibire a discarica - come è noto - presenta problematicità. Il Presidente della Regione, inoltre, potrà (questa è una modifica che abbiamo inserito in Commissione), in presenza di situazioni di criticità, definire con ordinanza i flussi dei conferimenti interprovinciali.

Sono iniziati i trasferimenti dei rifiuti verso la Puglia e verso l'Emilia-Romagna, mentre stanno per partire anche quelli destinati ad altre Regioni, tra cui il Lazio e la Toscana. Si tratta evidentemente di situazioni temporanee; temporanee; resta fermo, e deve restare fermo, il principio secondo il quale ogni ambito territoriale dovrà provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti. insomma ad avviare una normalità efficiente in Campania. In tale ottica, vanno lette tutte le modifiche apportate in Commissione e condivise dal Governo, che puntano ad un ulteriore snellimento ed accelerazione dell'*iter* per la costruzione degli impianti. Allo stesso obiettivo punta lo stanziamento di 150 milioni di euro per la realizzazione di piccoli impianti - di tutti quegli impianti intermedi che sono necessari - e per dare il via ad un programma che possa finalmente vedere una percentuale significativa di raccolta differenziata, che io ritengo la vera chiave di volta del problema dei rifiuti nel nostro Paese. Con una raccolta differenziata attestata a percentuali europee ed è questo un traguardo possibile anche in Campania, perché sappiamo che vi sono delle Province dove già oggi la raccolta differenziata è a livelli importanti si riduce in maniera significativa la quantità dei rifiuti da smaltire e che va trattata negli impianti di termovalorizzazione. Noi puntiamo anche ad una normalità condivisa. condivisa. La soluzione del problema dei rifiuti non può passare, com'è accaduto finora, attraverso una conflittualità continua tra le istituzioni del territorio. Io credo che la riattribuzione alla Regione di un ruolo di regìa forte

per i quali sono stati previsti requisiti di professionalità e di competenza per la realizzazione degli impianti ritenuti strategici. Alle Province è stata attribuita, in linea con quanto è stato previsto dalla Giunta regionale della Campania con due leggi (del 2007 e del 2008), la competenza ordinaria sui rifiuti, questa, che è stata letta in chiave politica e strumentale. Ciò che il Governo ha fatto è stato invece confermare una scelta che era stata assunta dalle istituzioni campane, all'epoca peraltro guidate dal centrosinistra. Si tratta tuttavia di un potere che era e che resta nella potestà della Regione, che potrà mutare l'indirizzo, se lo riterrà opportuno, ed individuare una modalità diversa. Noi non abbiamo inteso in alcun modo penalizzare i Comuni, e in questa ottica abbiamo recepito le proposte di entrambi gli schieramenti, disponendo una proroga di 12 mesi nel passaggio delle competenze dai Comuni alle Province e, quindi, il mantenimento in capo ai Comuni del diritto di riscossione della tassa sui rifiuti fino al 31 dicembre 2011. L'obiettivo di questo decreto, quindi, non è di dividere o di creare frizioni tra le istituzioni locali, ma semplicemente quello di aiutare e di assistere la Campania nel superamento di tutti i ritardi accumulati, cercando di avviarla nel più breve tempo possibile verso un regime virtuoso di trattamento e smaltimento dei rifiuti, in un sistema di collaborazione tra le diverse competenze locali e lo Stato. Io penso che questo obiettivo sia stato raggiunto, anche grazie al confronto costruttivo che si è svolto in Commissione, prima alla Camera e poi anche qui al Senato. Tale confronto ha consentito anche di aggiungere al provvedimento misure che io ritengo di assoluto rilievo sul fronte della civiltà e della legalità, in una Regione in cui purtroppo il settore dei rifiuti risente di pesantissime infiltrazioni da parte delle ecomafie. Mi riferisco alla norma, che abbiamo reintrodotto in Commissione, che prevede sanzioni penali per l'abbandono dei rifiuti. Tali norme erano state previste nel decreto del 2008 ed erano venute meno con la chiusura della fase emergenziale; noi le abbiamo qui prorogate, perché hanno prodotto dei risultati significativi. Concludo ribadendo la soddisfazione per il lavoro svolto, ringraziando tutti i senatori e tutte le senatrici per i contributi forniti in Commissione e per quelli che verranno in Aula. Sono convinta che abbiamo fatto davvero un buon lavoro per l'ambiente e per la Campania.

il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. Esaminati altresì i relativi emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri: sull'emendamento 1-*bis*.0.6 parere non ostativo, osservando che la norma, quanto alla individuazione puntuale dei siti di discarica, appare di eccessivo dettaglio ed è quindi suscettibile di ledere l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni; sull'emendamento 3.2 parere non ostativo, rilevando che la disposizione, nella parte in cui individua puntualmente le percentuali di ripartizione dei fondi, appare eccessivamente dettagliata e, conseguentemente, lesiva dell'autonomia regionale; sull'emendamento 3.0.1 parere non ostativo, invitando a specificare, al comma 1, se l'intesa ivi prevista debba aver luogo esclusivamente con le Regioni interessate ovvero se debba avere un carattere generale; in tal caso, sarebbe necessario il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni; - parere non ostativo sui restanti emendamenti». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto dei chiarimenti dei Governo sull'articolo 1, comma 7, e sull'articolo 2, comma 1, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo richiamando, tuttavia, l'attenzione del Governo al rispetto più puntuale dei criteri di costruzione del bilancio a legislazione vigente, secondo cui ogni innovazione legislativa deve essere corredata di nuove risorse di copertura. Il parere non ostativo sull'articolo 1, comma 7, è reso nel presupposto che gli eventuali maggiori oneri saranno coperti attraverso un incremento della tariffa

con prevedibili riflessi sul fabbisogno, il Governo dovrebbe fornire elementi di quantificazione più precisi». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.2, 1.380, 1.100, 1.5, 1.37, 1.41 (testo 2),

sulla proposta 3.101. Esprime poi parere non ostativo reso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti condizioni: che alla proposta 1.18 (testo 2) le parole: "con oneri quantificati in euro 350 mila a valere sulle risorse di cui al successivo articolo 3, comma 1" siano sostituite dalle seguenti: "alle spese di funzionamento della struttura di supporto si provvede nel limite massimo di euro 350 mila nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1". Sulla medesima proposta, analogamente a quanto osservato sul testo, la Commissione osserva infine che il Governo dovrebbe fornire elementi di quantificazione più precisi sull'analisi degli effetti finanziari delle norme sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di disposizioni aventi l'effetto di accelerare il profilo della cassa con prevedibili riflessi sul fabbisogno; che alla proposta 1.40 (testo 2) dopo la parola: "provvede" siano aggiunte le altre: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente incluse quelle indicate all'articolo che alle proposte l-*bis*.0.100 e 3.0.100, al primo periodo, siano aggiunte le seguenti parole: "fermo restando l'obbligo di garantire, con oneri a carico dell'utenza, l'integrale copertura dei costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti".

appare sproporzionata ed iniqua, anche perché il Comune di Camigliano, per le tante iniziative sui progetti di salvaguardia ambientale, entra addirittura nell'elenco dei Comuni virtuosi.

nel nuovo contesto normativo, di revocare per sopraggiunte ragioni di interesse pubblico il decreto di rimozione del sindaco e di scioglimento del comune di Camigliano e di reintegrare il sindaco nella sua funzione. Credo che sarebbe veramente un atto di giustizia.

di duplice denuncia. Intanto, segnalare il carattere propagandistico dell'approccio che il Governo ha seguito in questi quasi tre anni nella gestione legislativa e anche amministrativa di questo problema. denunciare il fallimento di questo approccio. Ho ascoltato con attenzione e anche con speranza l'intervento della ministro Prestigiacomo. Con speranza, perché, a oltre a oltre due anni e mezzo dal giorno in cui il presidente del Consiglio Berlusconi disse che nel giro di una settimana il problema dei rifiuti in Campania sarebbe stato risolto e di fronte all'evidenza (che tutti possono constatare) che mi auguravo che la ministro Prestigiacomo avrebbe avuto almeno il buon senso di riconoscere che qualcosa non ha funzionato nella scelta di puntare tutto sulla propaganda e anche nell'articolazione delle risposte al problema dell'emergenza rifiuti in Campania. Purtroppo la mie speranze sono andate deluse perché la Ministro, o il Ministro, Il ministro Prestigiacomo ha ripetuto la solita storiella che ci sentiamo ripetere da più di due anni e mezzo, e cioè che sostanzialmente siamo tornati alla normalità

confermano. Quindi, confermano che il Governo e la maggioranza proseguono con una strategia che mi dispiace definire dell'inganno dell'inganno dei cittadini, di chi magari non abita in Campania e non può direttamente vedere qual è la situazione e - fatto ancor più grave - dei cittadini campani che pagano sulla loro pelle la mancata soluzione

se le colpe di quello che non va sono dei Comuni, anche i meriti di quello che va sono dei Comuni. Mi riferisco, ad esempio, al merito dei tre Comuni campani superiori ai 20.000 abitanti che hanno

dell'approccio ingannatorio e propagandistico del Governo e della maggioranza. Infatti, dopo essersi presentato al Paese, quasi tre anni fa, dicendo che in pochi giorni tutto sarebbe stato risolto e sarebbero stati chiusi 16 anni di gestione straordinaria dei rifiuti; dopo aver formalmente chiuso la gestione commissariale, che è scaduta il 31 dicembre 2009, dando per risolto un problema che oggi è forse ancora più incancrenito di quanto non fosse a suo tempo,

nell'amministrazione e nella gestione del ciclo dei rifiuti in Campania, attraverso deroghe all'ordinaria amministrazione, deroghe all'ordinaria legislazione, deroghe all'ordinaria giurisdizione. Anche in questo decreto-legge le deroghe sono innumerevoli. Cito soltanto le principali, quelle più significative: all'articolo 1, comma 2, si prevede che il presidente della Regione possa nominare dei commissari straordinari, i quali, in virtù di un emendamento presentato al Senato dal relatore, si vedono attribuiti in maniera esplicita gli stessi poteri che fino a qualche mese fa aveva il sottosegretario Bertolaso;

transitorio di un anno, si conferma la scelta profondamente sbagliata di assegnare alle società provinciali non solo la gestione del ciclo dei rifiuti, ma anche la riscossione della TIA e della TARSU, ossia della tariffa o, a seconda dei casi, della tassa sullo smaltimento dei rifiuti. In questo modo si commette un'ingiustizia

attestati sugli standard migliori delle Regioni del Nord del Paese. Vi è poi un'altra deroga, sempre all'articolo 1, comma 2, dove vengono ridotti della metà i termini per le autorizzazioni, per le certificazioni, per i nulla osta in capo ai commissari straordinari, e dove si introducono e consolidano eccezioni per quanto riguarda il parere di valutazione di impatto ambientale. Ulteriori peggioramenti sono stati introdotti al Senato: come ho già

ingannatorio. Non si ha il coraggio di ammettere che non si è stati capaci di affrontare, e tanto meno di risolvere, l'emergenza, e si continua a non chiamare l'emergenza con il suo nome. Per questa ragione, abbiamo presentato l'emendamento 1.1, sfidandovi se non altro a chiamare le cose con il loro nome. O siete capaci di affrontare l'emergenza senza scaricarne le colpe soltanto sui vostri avversari politici o, se non altro, abbiate il buon senso e il buon gusto di chiamarla con il suo nome!

vicino al realizzando nuovo policlinico di Caserta. Dunque, veramente un contrasto tra salute e non salute.

infatti, che non si tratta di fare riferimento ad altre Regioni, ma per evidenti motivi di opportunità sarebbe rilevante inserire nella norma questo tipo di definizione.

colleghi, come ricordava la collega, il testo prevede che possano essere nominati commissari soltanto appartenenti alla carriera prefettizia, avvocati dello Stato e magistrati; a questi si aggiungono professori universitari con specifiche competenze tecniche. Mi pare obiettivamente difficile immaginare di avere criteri così stringenti e inoltre, una norma che in base all'eventuale militanza politica - che peraltro per questi soggetti mal si concilia con gli incarichi sul territorio

in quanto non è detto che una persona che ricopre ruoli universitari e ha competenze specifiche non abbia potuto svolgere un incarico politico istituzionale. Accade in Campania

l'emendamento 1.19 fa riferimento a quelle aree messe a disposizione dalle Province per lo smaltimento; quelle Province che hanno già dato una fortissima disponibilità, ferma restando la produzione dei rifiuti che fa riferimento alla Provincia stessa. Credo questo rappresenti anche un momento di equilibrio e di compensazione dove ognuno si assume una responsabilità rispetto alla produzione dei rifiuti e al completamento del ciclo integrato degli

parlare per dichiarazione di voto. che un quadro di leale e seria collaborazione fra tutte le istituzioni pubbliche interessate sia la base per delle scelte razionali e condivise. nella fase di progettazione e costruzione dei termovalorizzatori sia riconosciuto anche ai Comuni nel cui territorio ricadranno gli impianti un ruolo attivo, attraverso il meccanismo dell'intesa con il commissario straordinario nominato dal presidente della giunta regionale.

comunità sono contrarie), che i Comuni partecipino attivamente alla fase della progettazione e della costruzione, perché il loro ruolo è indispensabile e funzionale alla risoluzione del problema.

Ora, non è stato assolutamente piacevole vivere questa emergenza e continuarla a vivere, anche se in modo diverso. Vede, signor Ministro, se lei fa una passeggiata

Voglio fare un altro esempio. Il passaggio di tutta la riscossione delle tasse alle Province, la cosiddetta provincializzazione, signor Ministro, benché abbiate proposto un differimento dei termini, produrrà molto probabilmente un disastro. Si parla di federalismo municipale e decidiamo che la riscossione dei rifiuti venga fatta dalle Province?

Immaginate quando le Province dovranno riscuotere questi, di tributi, immaginate il tempo che ci vorrà per passare i ruoli, per informatizzare gli uffici, per produrre strumenti di controllo e di riscossione certa. Come faranno le Province, le Province da voi amministrate in questo momento? Come faranno a trovarsi esposte sul fronte delle tasse che non riscuotono, delle spese per la società, dell'assorbimento del personale? Ma vi rendete conto di quale mostro state producendo? Ad un certo punto vi ritroverete di nuovo qui, con un altro decreto, a chiederci di riprorogare dei termini, o magari vi renderete conto che alcune scelte erano sbagliate

tempo necessario per realizzare un termovalorizzatore degno di questo nome. È questo che ci preoccupa, signor Ministro. Ci preoccupano il tipo di procedura, le modalità

allora il coraggio di dire che l'emergenza c'è ancora e che occorrono dei poteri straordinari e abbiate il coraggio di lavorare in tal senso. Ma non utilizzate questo, come avete fatto, per dire di aver risolto una situazione, che - ci creda

Informo i colleghi che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti del Liceo ginnasio «Ugo Foscolo» di Albano Laziale, in provincia di Roma, ai quali diamo il benvenuto.

di trasparenza e di concorrenza, assicurando che sia esperita una gara. Come abbiamo detto questa mattina in Aula, sappiamo quanta delinquenza e quanta camorra c'è vicino a queste cose.

che il parere contrario su questo emendamento, come abbiamo già spiegato in Commissione, dipende dal fatto che il rispetto della normativa comunitaria è doveroso, anche se non è scritto nella norma. È un obbligo comunque. è del tutto pleonastico, perché è interesse del Governo e della maggioranza che vi sia il massimo rispetto della legalità, in particolar modo con riferimento a procedure di questo tipo. Quindi, è come se fosse stato accolto. Non è assolutamente

diamo la possibilità al Governo di utilizzare delle cave, se le norme lo consentono, ma per far sì che si trovino poi delle discariche. Visto che è possibile, approviamo l'emendamento; non capisco perché alla fine

scrivania. In detta ordinanza, signora Presidente, all'articolo 20 si costituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura nell'ambito del Segretariato generale della medesima. Le chiedo, della medesima. Le chiedo, signor Ministro, di prestare cortesemente attenzione: credo che non la conosca. Le finalità di questa nuova struttura sono di assicurare funzionalità e celerità ai processi decisionali in materia di gestione delle attuali criticità inerenti al ciclo integrato dei rifiuti nella Regione Campania, in sinergia con le amministrazioni territoriali interessate. Cosa significa questo? Siamo in presenza di un fatto estremamente singolare (dire irrituale è poco): negli stessi giorni, l'11 novembre 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri emana un'ordinanza di protezione civile con la quale, fra le altre cose, nomina una struttura con queste finalità espressamente delegata ad intervenire sui rifiuti in Campania; 16 giorni dopo, il 26 novembre 2010, lo stesso Presidente del Consiglio, insieme a tutto il Governo, approva il decreto-legge che stiamo esaminando. Qui si creano automaticamente e oggettivamente elementi di contrasto di poteri di livelli contrapposti. Non si riesce a capire a cosa serva. Ci sono alcune interpretazioni: una potrebbe essere quella, di fronte alla possibilità - come diceva la collega Incostante poco fa - del fallimento quasi certo di questo decreto, di tenere nella riserva appunto gli interventi derogatori della Protezione civile per reintervenire, anche se la Protezione civile è decaduta nei suoi poteri in materia di rifiuti a Napoli a fine 2009, con un bilancio tutto sommato estremamente negativo; l'altra, molto più vicina alla verità, è forse il sovrapporsi di diversi livelli, la mancanza di comunicazione fra i vari livelli della pubblica amministrazione e dei e dei membri di questo Governo, anche se entrambi questi provvedimenti legislativi sono firmati dalla stessa persona, il presidente Berlusconi (però un po' di distrazione di questi tempi è concessa). Credo che l'onerosità e l'irragionevolezza di questa ordinanza si capiscano fondamentalmente come necessità di allocare in altro posto gli ideologi e i grandi pensatori che hanno portato al *flop* della società Protezione civile S.p.A. Infatti, negli stessi giorni, il 10 novembre 2009, è stata presentata un'altra ordinanza

nel testo, prevedendosi con una norma che, attraverso società provinciali, la Provincia stessa gestisca gli impianti, affermandosi così una provincializzazione della gestione del ciclo integrato dei rifiuti che non è coerente con il resto della legislazione d'Italia. Si va sempre più verso una compressione insopportabile del ruolo dei Comuni e una confusione rispetto al ruolo delle Province, perché le Province hanno una funzione di controllo e pianificazione, mentre in Campania, in maniera del tutto anomala, avrebbero la gestione degli impianti, la gestione dei consorzi e la riscossione addirittura della TARSU e della TIA,

Presidente, signora Ministro, noi stiamo discutendo, come i colleghi hanno più volte ribadito, un decreto nel quale voi vi rifiutate di dichiarare che l'emergenza ci sia ancora.

In questo caso, ci permettiamo di esprimere un suggerimento di buon senso, cioè prevedere che si possano utilizzare

al relatore e al Governo perché vogliano esaminare la possibilità di esprimere parere favorevole su questo emendamento e di accogliere una proposta che è, appunto, di buon senso.

abbiamo presentato l'emendamento 1.34 per una ragione di coerenza con quanto fatto, o con quanto non fatto, o con quanto non ancora fatto, e per una ragione oggettiva anche di linearità rispetto al provvedimento in esame. L'impianto complessivo del decreto, come tanti colleghi fino a questo momento hanno avuto modo di evidenziare, viaggia su tutt'altra lunghezza d'onda. A me pare, francamente, che questa iniziativa a due velocità non sia congrua, ma sia piuttosto strana. Per questa ragione, il parere contrario del relatore e del Governo rispetto a questo emendamento mi sembra una inutile negazione dell'evidenza. Il problema non è ancora risolto, e lo sappiamo bene - chi più, chi meno - noi che viviamo nei territori della Campania.

la collega Armato ad altro proposito, potrei parlare della caparbietà con la quale il Governo continua a gravare le Province di competenze che per attitudini, oltre che per dimensioni istituzionali e territoriali, esse non sono in grado di ricoprire,

ad un ritorno all'ordinario, ma non ci sono al momento le condizioni, salvo che non si voglia concepire una norma che sancisca quanto di fatto e sostanzialmente non si è ancora verificato, ma che noi auspichiamo si verifichi

di trasferire oltre i confini regionali, e forse nazionali, i rifiuti della Campania, ciò significa - questo almeno è il segnale più evidente - che quell'emergenza non è finita.

parere contrario

il Governo preferirebbe la riformulazione del relatore subordinatamente al parere della Commissione bilancio,

Prevediamo, ad esempio, 50 milioni di euro per la realizzazione, il completamento o l'acquisto da parte di gestori del ciclo dei rifiuti di impianti di supporto al ciclo di valorizzazione delle raccolte differenziate. Ci proponiamo inoltre di operare nel campo della costruzione di impianti di compostaggio della frazione organica di rifiuti urbani, e di stanziare 100 milioni di euro per lo sviluppo delle raccolte differenziate, dando priorità ai sistemi domiciliari per la raccolta degli imballaggi

maggiori risorse a disposizione, riuscirebbero non soltanto ad inculcare nella cittadinanza un approccio differente nella gestione del rifiuto, e culturalmente mutato rispetto ai troppi vizi del passato,

rappresenta anche un modo di guardare al futuro con una certa lungimiranza, cercando di prevenire i problemi prima che si verifichino, e quindi anche dal punto di vista finanziario, prevedendo risorse adeguate per farvi fronte in modo tale che non si ripropongano in futuro. [DELLA

L'ordine del giorno reca la votazione per l'elezione di nove componenti effettivi e nove componenti supplenti della delegazione presso le Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa e dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO). A norma dell'articolo II della Carta dell'Assemblea parlamentare dell'UEO, i componenti della delegazione presso tale Assemblea sono infatti gli stessi che compongono la delegazione presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Nella presente circostanza, al rinnovo si procede mediante votazione in Assemblea, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento. Un'unica votazione a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento, avrà ad oggetto le seguenti liste predisposte in base alle designazioni dei Gruppi parlamentari: Componenti effettivi, senatori: Nessa, Santini, Saro, Valentino, Bricolo, Chiti, Giaretta, Marcenaro, Bugnano. Componenti supplenti, senatori: Ciarrapico, Balboni, Dell'Utri, Tofani, Boldi, Carloni, Crisafulli, Soliani, Carlino. Passiamo quindi alla votazione. I senatori favorevoli alle liste proposte voteranno sì. I senatori contrari voteranno no. I senatori che intendono astenersi si comporteranno di conseguenza. Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, sulle liste di cui si è data lettura. *(Segue la votazione)*

Proclamo pertanto eletti come componenti effettivi i senatori: Nessa, Santini, Saro, Valentino, Bricolo, Chiti, Giaretta, Marcenaro, Bugnano; e come componenti supplenti i senatori: Ciarrapico, Balboni, Dell'Utri, Tofani, link apre una nuova finestra"). Comunico altresì che, d'intesa con la Camera dei deputati, la delegazione è convocata per giovedì 20 gennaio, alle ore 8,30, nella sede di Palazzo Valdina, per procedere alla propria costituzione, che ha luogo mediante 1'elezione di due distinti Uffici di Presidenza, uno riferito all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e 1'altro riferito all'Assemblea parlamentare della UEO. Ricordo infine che alle relative votazioni potranno partecipare soltanto i componenti effettivi della delegazione e che solo questi ultimi potranno assumere cariche in seno agli Uffici di Presidenza, dovendosi limitare il ruolo dei componenti supplenti alla sola ipotesi di sostituzione dei titolari in caso di assenza o di impedimento.

vorrei cominciare questo mio intervento constatando una singolare circostanza che riguarda il provvedimento in esame oggi. È uno di quei decreti-legge, una minoranza in questa fase della storia parlamentare, a possedere i requisiti richiesti per la decretazione d'urgenza. È paradossale, però, il fatto che l'urgenza di questo decreto derivi in realtà non da una emergenza contingente, bensì da un fatto ormai strutturale, da quello che ormai è un dato fisso, che da quasi venti anni produce interventi e provvedimenti d'urgenza come questo.

Ancora una volta ci troviamo di fronte a un decreto-legge prodotto dall'immobilismo sul tema dei rifiuti in Campania. Un immobilismo che ha fatto dell'emergenza rifiuti di Napoli una potenziale fabbrica di decreti-legge d'urgenza a ripetizione; decreti con interventi anche importanti, come in questo caso, forse essenziali a tamponare le falle che si aprono periodicamente. In mancanza però di veri interventi strutturali e incisivi, questi decreti rischiano di diventare un rito di perpetuazione dello *status quo*. I primi interventi d'urgenza avevano avuto tra gli altri il merito di riaccendere la speranza verso una soluzione definitiva del problema; oggi i cittadini sono ormai sfiduciati. È comprensibile che di fronte a decreti che aprono nuove discariche o aumentano *ope legis* la capacità di quelle esistenti, in spregio alle esigenze dell'ambiente, del decoro del territorio e della tutela della salute, la speranza dei cittadini si tramuti in indignazione per poi sfociare in manifestazioni di rabbia (una discarica in particolare, quella di Cava Vitiello, sarebbe stata situata addirittura nel Parco nazionale del Vesuvio). Finché non si risolveranno i nodi di fondo la situazione non potrà che peggiorare. In questi ultimi anni, nella fase più acuta dell'emergenza, abbiamo assistito di continuo al varo di misure di urgenza: decreti-legge, interventi della Protezione civile e dell'Esercito, accompagnati da deroghe a disposizioni normative igienico-sanitarie, ambientali, sull'urbanistica e sul lavoro. Tutto per rattoppare ogni volta la falla di turno, rincorrendo sempre l'evolvere in peggio di un'emergenza ormai cronica, e per placare le manifestazioni sempre più diffuse e gravi di protesta dei paesi vesuviani i cui territori sono interessati dalle discariche. Questa impostazione emergenziale e commissariale non ha prodotto nulla. È stata proprio la Commissione europea a dirci che pur dopo venti anni di interventi urgenti e di commissariamento siamo di fatto all'anno zero per quanto riguarda i rifiuti di Campania. Non possiamo nemmeno ricominciare da tre, per citare un compianto attore napoletano: dobbiamo ricominciare da zero. È come se nulla si fosse mosso in questi venti anni. Non dimentichiamo che il 22 novembre 2010 Napoli è stata visitata dagli ispettori dell'Unione europea, i quali hanno svolto un sopralluogo per verificare lo stato di attuazione delle direttive in materia di gestione e smaltimento di rifiuti. Essi hanno constatato quanto poco sia stato fatto per risolvere alla radica il problema a tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Per di più, il piano regionale per la gestione dei rifiuti in Campania, al 31 dicembre 2010, non era ancora pervenuto alla Commissione europea. Ciò dimostra come la criticità della situazione investa vari livelli. Se ci saranno ulteriori ritardi nell'adeguamento per quanto riguarda la raccolta differenziata e la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti residui sarà impossibile sia rivedere la procedura di infrazione contestata dalla Corte di giustizia di Lussemburgo, sia sbloccare i 145 milioni di euro di fondi FAS destinati dal Governo alla Campania. Quando potremo finalmente vedere realizzato in Campania un ciclo integrale autosufficiente nello smaltimento dei rifiuti? La situazione in questi anni si è fatta cronica, certamente per le lentezze, i ritardi, le omissioni della Regione e del Comune di Napoli. Ma non dimentichiamo che in questi venti anni, forse anche più, nel territorio della Campania si sono riversati rifiuti provenienti da tutta Italia. *(Brusìo).* Presidente, non pretendo che mi si ascolti (lo dico anche a coloro

Ma non dimentichiamo che in questi venti anni, forse anche più, nel territorio della Campania si sono riversati rifiuti provenienti da tutta Italia. Individui senza scrupoli, delle regioni più ricche del Paese, hanno approfittato della situazione, e con l'aiuto delle ecomafie hanno fatto sparire tonnellate e tonnellate di rifiuti industriali che avrebbero dovuto altrimenti smaltire attraverso procedimenti costosi. In molti hanno tratto profitto dalla situazione di generale difficoltà sociale e istituzionale della Campania, della quale l'emergenza rifiuti è una delle manifestazioni. Hanno tratto profitto a spese del territorio, degli abitanti, delle bellezze e dell'immagine internazionale di Napoli e dell'Italia. Ma vi è di più. La Campania è la punta dell'*iceberg* di un'emergenza che, in assenza di volontà politica e di interventi veri e strutturali, rischia di estendersi ad altri territori del Paese, con costi incalcolabili per l'economia, l'ambiente e la salute. E allora le scelte devono essere fatte subito! Dobbiamo essere coscienti del fatto che proprio le normative comunitarie indicano un percorso preciso e obbligato per conseguire soluzioni strutturali al problema dei rifiuti, in termini di impiantistica e di raccolta differenziata. Si è parlato della costruzione di nuovi termovalorizzatori in Campania. Dobbiamo però essere realisti. Per realizzare materialmente nuovi impianti occorrono anni, se si includono anche i tempi per bandire la gara e relativo svolgimento per l'aggiudicazione. Questo decreto-legge assegna circa 150 milioni di euro di fondi FAS alla Campania per gestire e coordinare il ciclo dei rifiuti; dà la possibilità al Governo regionale di sostituirsi agli enti inadempienti, soprattutto in tema di incremento della raccolta differenziata; riconosce ai prefetti la possibilità di diffidare i Comuni che si dimostrano inadempienti rispetto agli obiettivi minimi di raccolta differenziata, nonché di nominare commissari *ad acta*. Vista poi l'urgenza di individuare le aree nelle quali localizzare gli impianti di recupero, produzione e fornitura di energia dal trattamento dei rifiuti, al Presidente della Regione Campania è riconosciuto il potere, sentite le Province e gli enti locali interessati, di nominare commissari straordinari con il compito di individuare le aree in questione. Ai presidenti delle cinque Province è invece affidato il compito di istituire un tavolo di coordinamento per individuare una soluzione definitiva all'emergenza contingente. Soluzione che purtroppo non potrà che concretizzarsi in prima battuta nella individuazione di due megadiscariche da 250.000 mila tonnellate di rifiuti, da realizzare entro il 2011 e di altre discariche nella zona del Nolano e di Napoli nord di livello comprensoriale. La vera sfida si gioca però sul piano della raccolta differenziata. Solo se gli enti territoriali, *in primis* i Comuni, sapranno svolgere un'azione di sensibilizzazione dei cittadini nei confronti della raccolta differenziata, il problema dei rifiuti potrà avere una soluzione strutturale e definitiva. Il riciclo dei rifiuti, basato sull'utilizzo simultaneo e sinergico dell'impiantistica e dei sistemi di raccolta differenziata, è la vera rivoluzione copernicana. Troviamo positivo il fatto che oggi sia il Ministro dell'ambiente ad intervenire in Assemblea per il Governo e non invece, come è avvenuto in passato, il Sottosegretario alla protezione civile. Speriamo che questo sia un primo segnale, un presagio di buon auspicio per il superamento della cultura emergenziale. Dichiariamo dunque un voto favorevole al provvedimento, certi di mostrare ancora una volta agli italiani il nostro senso di responsabilità, coscienti del nostro dovere nei confronti del Paese. Nutriamo però ancora la speranza che si tratti veramente dell'ultimo decreto-ponte e che si apra finalmente una nuova strada verso una soluzione strutturale e definitiva del problema rifiuti a Napoli e in tutta la Campania.

Non so se i colleghi della maggioranza si sono resi conto che insieme agli emendamenti dell'opposizione hanno respinto una serie di direttive europee e principi consolidati della legislazione comunitaria ai quali tali emendamenti facevano riferimento. Di fatto, avete bocciato persino il richiamo a norme e principi del decreto legislativo n. 205 del 2010, che questo stesso Governo ha approvato nemmeno due mesi fa. Questo è davvero un paradosso, nel momento in cui si proclama il rientro nell'ordinario. Le norme proposte, infatti, ignorano alcuni temi essenziali che abbiamo sollevato in discussione generale, evitano accuratamente di affrontare i nodi strutturali e non fanno intravedere, né la propongono, alcuna vera strategia di uscita a lungo termine dalla crisi. Venute meno le discariche previste dal precedente decreto‑legge 23 maggio 2008 n. 90, la soluzione principale a breve termine individuata dal Governo è sostanzialmente quella di chiedere solidarietà alle altre Regioni affinché ospitino i rifiuti campani e l'utilizzo delle cave dismesse. Del sistema di tracciabilità, delle ecoballe, della raccolta domiciliare obbligatoria, degli impianti di compostaggio e riciclo totale dei prodotti non c'è alcuna traccia. Resta intatto il collo di bottiglia. Nella corretta gestione del ciclo dei rifiuti, la provincializzazione dei medesimi ha penalizzato assolutamente anche i Comuni più virtuosi nella raccolta differenziata (e ce lo siamo detti diverse volte). Resta intatta anche l'incertezza sugli impianti di termovalorizzazione, sui quali ci si attarda a puntare e a dividersi: non solo si dovrà attendere molto tempo prima del loro pieno funzionamento, ma saranno inevitabilmente necessarie nuove discariche di stoccaggio. Quello che concretamente manca nel decreto sono le infrastrutture e gli impianti che consentano di gestire la fase intermedia dei rifiuti. In stretto raccordo con una politica di forte impulso alla differenziata, sarebbe indispensabile finanziare e semplificare la realizzazione di impianti per trattare l'organico, che consentono tra l'altro di ridurre drasticamente la quantità di rifiuti destinati alla discarica. In questi anni non si sono voluti realizzare i necessari siti di compostaggio, l'unico mezzo cosa che, eliminando la frazione umida, impedisce la fermentazione dei rifiuti in discarica, cosa assai grave visto che al Sud la frazione organica arriva al 50 per cento di tutta la differenziata. I rifiuti organici vengono invece portati in altre Regioni, arrivando a pagare fino a 200 euro a tonnellata per questo servizio. Inoltre, a differenza dei termovalorizzatori, gli impianti di compostaggio costano molto meno ed hanno tempi di realizzazione molto più rapidi. Ma, evidentemente, nessuno pensa di fare decreti-legge per rilanciare queste strutture e quelle per il riciclo totale dei cosiddetti rifiuti. Preferite invece derogare ancora una volta alla valutazione di impatto ambientale, alla certificazione pubblica, agli obblighi comunitari di gare d'appalto pubbliche (per affidare le opere con trattativa privata). Solo con gli interventi che trascurate, concretizzabili in meno meno di due anni, e con lo sviluppo di politiche di riduzione a monte degli imballaggi e dei rifiuti, si darebbe una soluzione di buona parte dell'emergenza in Campania, costata inutilmente agli italiani e ai campani in particolare, che pagano le tariffe più alte d'Italia, più di 3 miliardi di euro in 15 anni. Abbiamo proposto la chiusura della discarica «Cava Sari» nel Comune di Terzigno fino all'approvazione definitiva del nuovo piano regionale dei rifiuti conforme ai pertinenti obblighi derivanti dagli indirizzi dell'Unione europea in materia ambientale, degli indispensabili interventi di bonifica, nonché delle risultanze relative ai controlli ambientali e sanitari nel territorio circostante. In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui la discarica di Terzigno continui ad essere attiva, abbiamo ritenuto indispensabile, viste le condizioni sanitarie ed ambientali in cui versa la discarica, che sia autorizzato esclusivamente il conferimento della frazione secca dei rifiuti. Sui rifiuti pericolosi abbiamo proposto l'abrogazione della disposizione contenuta nell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. in nome dell'emergenza rifiuti, consente di poter conferire nelle discariche campane anche i rifiuti pericolosi (ceneri pesanti, fanghi con sostanze pericolose, eccetera). Dopo due anni e mezzo, visto che voi stessi avete dichiarato che è terminata l'emergenza vera e propria, è inaccettabile consentire di continuare a sversare nelle discariche anche i rifiuti pericolosi. È semplicemente illogico che, in nome di un'emergenza ambientale, si rischi un'emergenza sanitaria. Queste assurdità sono la causa dell'esasperazione della popolazione costretta a vivere in prossimità di discariche, visto che i cittadini non sanno cosa esattamente finisce in quelle aree. È per questo che abbiamo chiesto il superamento del continuo regime di deroghe. Ricordiamo che la statalizzazione, prima, e la provincializzazione, poi, dei rifiuti hanno finora rappresentato uno dei principali ostacoli al superamento delle continue emergenze rifiuti della Regione. Abbiamo perciò chiesto il mantenimento in capo ai Comuni - come avviene in tutti i Comuni d'Italia - delle attività di gestione dei rifiuti, ben oltre la semplice proroga di un anno della norma contenuta nel decreto‑legge n. 195 del 2009. vale anche per la gestione e la riscossione delle tariffe TARSU e TIA, che dal prossimo anno vengono invece assegnate alle Province. Abbiamo chiesto il rispetto della normativa comunitaria e, quindi, il rispetto della procedura VIA prevista dal codice ambientale per la realizzazione di tutti gli impianti, visto che l'emergenza - lo dite voi stessi - è finita. Il vantaggio di poter beneficiare di un risparmio di qualche settimana è molto minore del rischio di una procedura non accurata, visto che poi i danni durano per anni. Abbiamo chiesto controlli obbligatori sui rifiuti biostabilizzati utilizzati a copertura e risagomatura di cave abbandonate o dismesse e di discariche chiuse ed esaurite, ovvero quale materiale di copertura giornaliero delle discariche in esercizio, per verificare se effettivamente rispondono ai requisiti minimi richiesti. Va quindi vietata l'eventualità che il livellamento si faccia con il tal quale. Abbiamo chiesto un piano per la differenziata domiciliare e sanzioni per i Comuni inadempienti. L'Italia dei Valori è contraria al ricorso continuo a commissariamenti, tuttavia abbiamo proposto che i futuri commissari previsti dal decreto siano scelti sulla base delle loro competenze e diano garanzie di indipendenza da qualunque appartenenza o condizionamento politico, onde prevenire pressioni, condizionamenti ed infiltrazioni di interessi non trasparenti. Tutte queste proposte sono state respinte senza una motivazione adeguata. Onorevoli colleghi, nel quadro delle problematiche tecniche del testo, vorrei ricordarvi inoltre che il regime sanzionatorio speciale di cui all'emendamento 1.200 presenta chiaramente alcuni profili di dubbia costituzionalità: motivo ulteriore per il quale riteniamo che questo provvedimento rischia di creare più problemi di quanti pretenda di risolverne. Per tutti questi motivi, il voto del Gruppo Italia dei Valori non può essere che contrario.

avendo peraltro già sostenuto in discussione generale la posizione del mio Gruppo sull'opportunità di votare a favore del provvedimento Non si tratta certo di un provvedimento perfetto, molte sono le lacune e molte sono le cose che avremmo voluto diversamente esposte. la reale urgenza di provvedere a superare lo stato delle cose imponga un senso di responsabilità a chi in qualche modo ha il dovere di esprimere di esprimere una modalità con la quale lavorare. Lo strumento legislativo che è stato oggi discusso è dunque uno strumento che ha anche la

Credo che oggi il Governo non abbia alcun alibi: gli viene consegnato uno strumento per poter operare. Penso che sia necessario farlo presto e bene, e per questo ci assumiamo oggi questa responsabilità. Altrettanto chiara deve essere oggi la responsabilità di chi governa. Con questa chiarezza, ci sentiamo serenamente di poter dire

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, per l'ennesima volta in quest'Aula ci troviamo ad affrontare l'emergenza rifiuti nella Regione Campania. Per l'ennesima volta ci troviamo a porre rimedi ad una situazione in cancrena ormai da 17 anni e a sopperire alle mancanze e all'incapacità delle amministrazioni locali nella gestione del proprio territorio. mi riferisco soprattutto al Comune capoluogo di Regione, Napoli, e a quella parte politica e amministrativa che ha mandato in rovina l'economia, il turismo e l'immagine di questo territorio, ha compromesso i diritti fondamentali e la salute della popolazione, danneggiando anche l'immagine dell'intero Paese verso il mondo intero, perché la Campania è diventata ormai il paradigma che ha fatto il giro del mondo, a dimostrazione di che cosa porta una politica locale basata su clientelismi, sprechi e assunzioni spropositate e di comodo. Di certo non si tratta di inventare soluzioni nuove sulla gestione dei rifiuti. Basta guardare e imitare gli esempi eccellenti del Nord, della Lombardia e del Veneto, sulla valorizzazione dei rifiuti, il recupero dei sottoprodotti, la raccolta differenziata e la raccolta porta a porta. Oramai lo hanno capito tutti che qui si tratta di una vera volontà di mantenere in vita un'emergenza continua, speculando sulla qualità della vita dei cittadini e sprecando le risorse pubbliche, per perseguire interessi che non favoriscono altro che la criminalità organizzata collegata al ciclo dei rifiuti. L'opposizione, strumentalmente, vuole far ricadere le responsabilità sul Governo. Il nostro Governo, invece, è l'unico che, sin dall'avvio della legislatura, si è impegnato seriamente a risolvere l'emergenza rifiuti della Regione Campania. Il 31 dicembre 2009 si è conclusa una fase di emergenza che durava dal 1994 e proprio per la durata del periodo emergenziale ha richiesto interventi forti e complessi. Il provvedimento in esame non è altro che un correttivo dei provvedimenti di urgenza già emanati, che definisce e conclude un percorso tracciato dal Governo per ristabilire nella Regione la gestione ordinaria dei rifiuti, in linea con il resto del Paese e in linea con le norme europee. Si tratta di misure necessarie per poter consentire il subentro degli enti territoriali campani nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. che le soluzioni finanziarie si trovano direttamente all'interno delle risorse già assegnate alla regione Campania e questa volta attingono in particolare ai fondi FAS attribuiti a tale Regione, per 432 milioni di euro. Ciò serve anche per responsabilizzare la classe dirigente sulla necessità di chiudere al più presto una situazione dissennata, che manda letteralmente in discarica risorse che altrimenti sarebbero utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche. Altre amministrazioni locali, ovviamente più virtuose, riescono dalla tariffa o dalla tassa sui rifiuti, dal recupero dei sottoprodotti e dal riutilizzo dell'umido, a raggiungere un bilancio positivo della gestione del ciclo dei propri rifiuti, senza necessità di adoperare altre risorse finanziarie. Il Gruppo della Lega Nord Padania voterà a favore della conversione in legge del presente decreto, che non fa altro che confermare l'impianto già impostato due anni e mezzo fa dal nostro Governo, nell'obiettivo di consentire a Napoli e alla Campania di avviare al più presto un ciclo di smaltimento dei rifiuti moderno e in linea con quanto accade in altre parti del Paese e dell'Europa ed in particolare nei nostri territori padani. Il nostro voto va colto unitamente alla lucida consapevolezza che, se il senso di responsabilità civica - che auspichiamo possa tornare a contraddistinguere l'operato degli amministratori locali campani non trovasse empirica e concreta conferma nei fatti, il Paese intero, ed il Nord in particolare, non potrebbero certamente continuare a sopportare ulteriormente spese così pesanti per far fronte ad una emergenza che, contrariamente ad una fase di naturale temporaneità e provvisorietà,

Signor Presidente, egregi colleghi e colleghe, mi sia consentito partire da una constatazione:

se ci ritroviamo ad affrontare la questione dei rifiuti della Campania per la quinta volta, dobbiamo riflettere sul fatto che evidentemente i decreti legge finora predisposti e approvati, così come noi del Partito Democratico abbiamo fatto notare ogni volta con grande senso di responsabilità, non risolvevano e non possono risolvere questa questione. Non è certamente quest'ultimo decreto che elimina le storture che rischiano di alimentare altra confusione e perpetrare una situazione che è oramai ridicolo definire di emergenza. Ha ragione il collega Della Seta: bisogna avere coraggio e chiamare le cose per nome e cognome e far riferimento a un vero stato di emergenza, che oggi tocca la Campania e non so se nei prossimi mesi non toccherà anche altre Regioni del Mezzogiorno. Quando si dispone, come si fa in questo testo, che la titolarità della TARSU va sottratta ai Comuni e assegnata alle Province, anche se la Camera ne

resta attualissima l'analisi dell'ANCI che fa riferimento al decreto n. 195 del 2009 parlando di una transizione mancata per un'equilibrata e funzionale articolazione delle responsabilità e dei compiti tra istituzioni decentrate. Si profilano ulteriori megastrutture destinate ben presto a configurarsi come nuovi ed improduttivi carrozzoni, i cui costi comporteranno inasprimenti tariffari e pregiudicheranno le esperienze positive in atto in molti Comuni della Campania, producendo deresponsabilizzazioni e un livellamento verso il basso. I Comuni della Campania, nell'ambito della leale cooperazione tra istituzioni della Repubblica, non escludono il conferimento di ulteriori funzioni alle Province, purché ciò avvenga nel quadro di una strategia condivisa e complessiva, utile per i cittadini. Che fine ha fatto, chiedo al senatore Leoni e alla Lega Nord, il federalismo fiscale? non lo abbiamo relegato né dimenticato; e anche per evitare che sulle Province della Campania finisca col gravare un accumulo di criticità in termini di disservizi e costi, già evidente nella società provinciale costituita, chiediamo che la riscossione della TARSU torni definitivamente in capo ai Comuni. Il ritorno all'ordinario nella gestione del ciclo dei rifiuti passa attraverso la responsabilizzazione di tutti i livelli istituzionali, che devono svolgere ciascuno la propria parte per il bene della comunità. Il 18 luglio 2008, Berlusconi, battendo sulla grancassa della propaganda politica, secondo una sua abitudine, proclamò *urbi et orbi*: "Napoli è tornata in Occidente, in Campania lo Stato è tornato a fare lo Stato", annunciando che sarebbero bastati pochi mesi per uscire dell'emergenza. Tutto falso, tutte balle. A settembre dell'anno appena trascorso la crisi è tornata ai livelli drammatici del 2008 e annulla sono valse le promesse di Berlusconi, che ha giocato, senza successo, anche la carta del *jolly* Bertolaso. Tutto inutile: il nostro primo Ministro se ne dispiacerà, ma il primato dei miracoli a Napoli resta saldo nelle mani di San Gennaro. Intanto, il risultato della campagna pubblicitaria del centrodestra, cui fanno riferimento la Regione e quattro delle cinque Province della Campania, è che l'emergenza è ancora lì, la TARSU è tra le più alte d'Italia, le comunità sono pronte a dare battaglia per impedire che si aprano nuovi sversatoi e le discariche esistenti sono prossime all'esaurimento.

e gli impianti di complemento, quando e dove costruiti, si sono rivelati assolutamente inadeguati, per non dover dire che gli altri termovalorizzatori non sono ancora partiti. mentre i rifiuti della Campania vengono inviati in Puglia, in Emilia Romagna, nel Lazio (un compattatore al giorno) o in Calabria, per parlare di un'altra realtà in grave crisi, c'è da affrontare la questione, che è anche sociale, dei debiti lasciati dai consorzi in liquidazione. Per i dipendenti che aspettano lo stipendio e non hanno certezza alcuna sul loro futuro lavorativo, occorre un vero e proprio piano sociale del Governo che dovrebbe farsi carico di questa prospettiva. Intanto, sul territorio sono accatastati circa sette milioni di ecoballe, che di eco non hanno nulla e, anche se Berlusconi e i suoi uomini fingono di non saperlo o immaginano che possano essere dimenticate, continuano ad avvelenare l'ambiente già imbottito, specie nel napoletano e nel casertano, di rifiuti pericolosi giunti dalle industrie del Nord attraverso la premiata ditta «Camorra Spa». In Commissione di inchiesta sugli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti, il presidente della Regione, Stefano Caldoro, ha dichiarato che per archiviare la crisi occorrono da tre a quattro anni, denunciando in sostanza che l'emergenza non era finita profilando all'orizzonte il rischio di perdere i fondi stanziati dall'Unione europea e attualmente congelati, mentre il ministro dell'ambiente Stefania Prestigiacomo il 13 gennaio consegnava alla Commissione ambiente dati molto preoccupanti. «Occorrono nuovi siti», ha detto, ma nel decreto-legge che ci chiedono di approvare non figura alcuna indicazione in tal senso. Mi fa piacere che il ministro Prestigiacomo abbia accolto con maggiore senso di responsabilità e determinazione l'indicazione, già al centro dell'ordine del giorno approvato all'unanimità dal Senato il 9 luglio 2008, ad utilizzare le cave abbandonate o dismesse presenti in Campania e abbia deciso di inserirla nel testo della relazione al decreto-legge utilizzando tali siti, e non è una mia ostinazione, si centreranno tre obiettivi, rispondendo concretamente alle esigenze delle comunità, bonificando queste cave che sfregiano - vere e proprie artigliate nelle montagne - il panorama unico della nostra Regione, e assestando un duro colpo alla criminalità organizzata che, come risulta da inchieste ed indagini, detiene il monopolio sulla gestione di gran parte di tali aree, spesso utilizzate per sversarvi veleni industriali e rifiuti tossici. Il Governo potrebbe dare un segnale forte, avviando, come dicevo, l'opera di recupero ambientale del territorio, ancora al palo nonostante le risorse stanziate ed utilizzate dal Commissariato bonifiche, eppure straordinaria opportunità, anche per le ricadute occupazionali, di rinascita e sviluppo. Credo sia doveroso, anche per recuperare credibilità allo Stato e alle istituzioni, bonificare i territori in cui insistono i siti utilizzati per il deposito e il trattamento dei rifiuti, così come credo che sia fondamentale chiudere nel cassetto spot e proclami e avviare un piano strategico serio per definire tutti i passaggi, assegnando ruoli e responsabilità precise, in cui va articolata una gestione seria, responsabile e finalmente integrata dei ciclo dei rifiuti in Campania. Da Vice Presidente della Commissione di

La drammaticità della situazione ci impone una riflessione seria e responsabile e scelte strategiche scevre da tatticismi e tentazioni demagogico-propagandistiche.

potrebbero trovarsi a dover fare i conti con le stesse criticità, anche con maggiore drammaticità. Sta a noi raccogliere il grido di aiuto di queste comunità e far sentire, in maniera determinata, la presenza dello Stato

letteralmente violentato da una criminalità aggressiva, predatoria, che sul piano più generale dell'intero Paese - come ha rivelato Legambiente nell'ultimo rapporto - ha nella distruzione dell'ambiente, finalizzata al traffico di rifiuti, il 25 per cento del fatturato annuo. Riportare sui binari della legalità e dell'organizzazione integrata la gestione del ciclo dei rifiuti servirà anche ad eliminare l'assurda e pericolosa diseguaglianza tra il Nord e il Sud del Paese. lavorare per definire il percorso di rilancio della Campania, del Mezzogiorno e del Paese, offrendo un contributo positivo e costruttivo alla risoluzione della crisi dei rifiuti in Campania e nel Mezzogiorno, sulla quale sarebbe auspicabile andare oltre le casacche politiche. Ciononostante, il Governo continua ad indulgere alla demagogia, evitando di dare risposte responsabili e di prospettiva ad una crisi che è sociale, economica e democratica, la quale richiede interventi risolutori netti e radicali. esprimiamo, seppure con rammarico, un voto contrario a questo decreto che - a nostro avviso - perpetra la logica dell'emergenza senza una prospettiva di certezza e di civiltà per questo Paese.

approfittare dell'occasione per ringraziare tutti i senatori che hanno partecipato al dibattito, sia del nostro Gruppo che degli altri Gruppi parlamentari,

Non è propaganda che tutta una serie di interventi sia stata fatta anche per reperire nuovi siti e per inaugurare nuovi luoghi dove allocare i rifiuti È propaganda, ma in senso negativo, tutto ciò che accade nelle strade di Napoli quando i commissari straordinari - mi riferisco segnatamente al periodo del sottosegretario Bertolaso - individuavano nuovi siti e voi scatenavate la guerra nelle strade perché non li volevate. però, ci venite a dire che siete preoccupati perché non si trovano nuovi siti o perché non sono stati ancora individuati, o che siete contrari alla nomina dei commissari per individuarli. Ci chiedete la chiusura di alcune discariche, una delle quali il Ministro ha riconosciuto di poter chiudere, venendo incontro alle istanze vostre e anche di molti nostri colleghi, e nel frattempo, però, ci dite che noi non risolviamo il problema dei rifiuti. Il problema dei rifiuti in Campania - tutti lo abbiamo ricordato - è assai annoso, ma non corrisponde assolutamente al vero che dura da 17 anni in maniera eguale. Il picco della crisi dei rifiuti in Campania è stato raggiunto nel 2007 e agli inizi del 2008, quando ‑ allora io ero membro della Commissione ambiente all'opposizione ‑ vi trastullavate - ricordo le diatribe interne tra il Ministro e il Presidente della Commissione, entrambi campani - a rincorrervi sui siti da aprire o da chiudere e, nel frattempo, i cumuli dei rifiuti a Napoli crescevano.

un regime pacificatorio soprattutto degli scontri a livello locale. Non è corretto mettere i Comuni contro le Province, perché, se esiste una possibilità di incontro, questa deve essere riservata alla nuova

la vicenda dei rifiuti campani. Non è possibile pensare che lo Stato debba sempre intervenire. Non fa piacere a nessuno intervenire con norme straordinarie, con norme in delega, con la nomina di commissari. Non fa piacere a nessuno - ripeto - ma con grande senso di responsabilità, quando se ne rileva la necessità, lo si fa, e lo si fa sempre cercando di ottenere risultati positivi. Questo è il significato che ci accingiamo ad approvare oggi, e non vogliamo ripercorrere la tragedia di tutti i consorzi messi in liquidazione, del clientelismo che per anni avete alimentato nella Regione Campania e a Napoli. Non vogliamo assolutamente insistere su argomenti, quelli sì, di facile propaganda. Per noi la vera propaganda sono i fatti. Il nostro manifesto elettorale sono le strade che percorriamo e, quando ci saranno le elezioni e la Regione Campania avrà assunto la sua responsabilità anche in termini operativi, certamente non si potrà dire che a Napoli non è stato fatto nulla, perché se non fosse stato fatto nulla oggi voi sostenete - i rifiuti di Napoli avrebbero già travalicato i confini regionali, e forse nazionali, nell'accumulo. Voi stessi avete detto che a Napoli si producono 7.000 tonnellate di rifiuti al giorno che non si riescono ad eliminare. Ma chi è che non li riesce ad eliminare? non riesce eliminare i rifiuti che si producono. Andiamoci molto piano anche con l'enfatizzazione della raccolta differenziata, che è sicuramente utile, ma che la stessa normativa europea

di percentuali che sono tutte da verificare corrisponde direttamente a una rilevazione di diminuzione del prodotto rifiuto, che non avviene per un'improvvisa

lì diminuisce la produzione di rifiuti, ma aumenta in maniera esponenziale nei quartieri contigui, dove il cittadino può continuare a sversare in maniera indifferenziata.

che la possono rendere efficace, e utile anche per la produzione di energia. È per questo che in questo decreto-legge abbiamo inserito una norma per sbloccare quei termovalorizzatori che i livelli locali hanno contrastato fino ad ora. Si è resa Si è resa necessaria ulteriormente una norma per far sì che i termovalorizzazione si realizzino. Credo che, come Commissione ambiente, abbiamo il compito di affrontare la tematica dei rifiuti nella sua interezza, per dare a questa a questa incombenza, a questo importantissimo servizio nei confronti dei cittadini, delle direttive alle Regioni e agli enti locali che ne sono responsabili. Ciò, al

che le popolazioni, ad ogni tornata elettorale, ce ne hanno riconosciuto il merito effettivo, creando un'assoluta inversione di tendenza nella classe politica campana, che ha dato e continuerà a dare fiducia al centrodestra, perché noi parliamo con i fatti e voi invece usate soltanto propaganda sterile e sicuramente improduttiva.

è integrato con l'informativa del Ministro della difesa sulla morte di un soldato del contingente militare italiano in Afghanistan. Dopo l'intervento del ministro La Russa, che avrà luogo attorno alle ore 10,45, potranno intervenire i rappresentanti dei Gruppi per cinque minuti ciascuno.

una singolare protesta, ossia chiudere i municipi un giorno alla settimana, perché gli obiettivi del Patto di stabilità interno previsti dalle nuove normative di fatto impediscono loro di amministrare correttamente i servizi nei propri territori.

guarda indietro, di dover rispettare, dei parametri relativamente agli anni passati, in cui non c'era l'obbligo del Patto di stabilità. Dovrebbe recuperare nel 2011, e quindi avere un obiettivo di bilancio in positivo, oltre 680.000 euro. Stiamo parlando di un Comune che ha in totale un bilancio di 3 milioni euro. Potete quindi comprendere che ciò è impossibile, a meno che non si chiudano i servizi. In questo senso, spero che vi sia la possibilità di affrontare in modo serio il Patto di stabilità

*(PD)*. Signor Presidente, nella scorsa seduta il Senato ha approvato all'unanimità

*(PD)*. Signor Presidente, nella scorsa seduta il Senato ha approvato all'unanimità una risoluzione contro la persecuzione dei cristiani, per la libertà di religione ed in particolare per la libertà delle minoranze. È stato un atto molto importante che riguarda la difesa di diritti umani fondamentali. Nei giorni scorsi, un tribunale egiziano ha condannato a morte uno degli autori dei delitti nei quali hanno perso la vita delle persone di fede cristiana. Io penso che sia nostro dovere - e lo chiedo al Presidente del Senato - esprimere la nostra richiesta che nessuna esecuzione capitale avvenga e che in nessun modo l'iniziativa importante che noi abbiamo deliberato possa essere confusa con un'azione che viola i diritti umani fondamentali. Il fatto che lo facciamo noi, che ci siamo espressi chiaramente su questo tema, penso abbia un valore particolare e credo che su questo, per le posizioni che ha sempre assunto, l'Assemblea del Senato non possa che convenire. *(Applausi

l'Italia, in tutte le sue forze politiche, si è sempre espressa contro la pena di morte, in qualsiasi circostanza. I colpevoli devono stare in carcere e non essere

al Patto di stabilità in ordine a quei Comuni, in special modo alcuni Comuni veneti, che vengano a trovarsi nelle condizioni che il senatore Stradiotto ha descritto così bene. Sono sicura che in Commissione bilancio, che congiuntamente alla Commissione affari costituzionali esamina in sede referente il decreto-legge milleproroghe potrà esserci lo spazio per trovare una soluzione a questo specifico fronte di Comuni che si trovano in questa particolare condizione. E, quindi, non solo condividendo il grido di allarme lanciato dal senatore Stradiotto, ma probabilmente anche un percorso in Commissione che ci possa portare in modo unitario ad affrontare e risolvere questo problema, esprimo la nostra totale disponibilità e il nostro impegno in tal senso.